L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

la discussione generale di ieri ha fatto emergere in maniera inequivocabile ciò che già avevo esposto nel corso della relazione introduttiva; esistono una generale condivisione ed una sensibilità particolare nei confronti di questo provvedimento da parte di tutte le forze politiche che hanno contribuito in maniera attiva, grazie anche alla sapiente direzione della Presidente della Commissione d'inchiesta, prima firmataria del disegno

L'unico collega che ha manifestato un'apparente contrarietà al testo in generale è stato il senatore Giovanardi, al quale però non credo sia neanche necessario rispondere perché, a mio parere, una lettura attenta del provvedimento stesso consente di fugare tutti i suoi dubbi,

aver spiegato ieri in maniera esaustiva il motivo per il quale non c'è alcun pericolo che le pene nei confronti dell'autore delle diffamazioni a mezzo stampa In quella relazione si legge testualmente: «In questa direzione sembrerebbe si siano mossi gli inquirenti nelle rare occasioni, a cui si è fatto cenno, in cui taluni atti intimidatori sono stati qualificati come violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 336 tuttavia, come osservato nelle audizioni effettuate dalla Commissione, non consente di distinguere tra amministratore locale e altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e di cogliere la particolarità della figura dell'amministratore locale il quale, pur svolgendo

svolgendo delle funzioni amministrative al pari di altri pubblici ufficiali, assume il proprio ruolo in virtù dell'esplicazione del principio democratico». In buona sostanza, si dice che l'applicazione dell'articolo 336 del codice penale non sarebbe adeguata, in quanto si rivelerebbe inidonea a cogliere quel *quid *quid pluris* che distingue l'offesa all'amministratore locale da quella diretta ad un altro pubblico ufficiale. È per questo motivo che nel testo è stata introdotta la modifica dell'articolo 338, specificando - così come suggerito nel corso delle stesse audizioni - che deve essere contemplato anche il singolo componente, seguendo, peraltro, anche quella giurisprudenza (che è la più recente

l'articolo 338. È, quindi, corretta la specificazione che è stata operata in questo provvedimento con riferimento all'articolo 338 del codice penale e non all'articolo 336, come auspicato dal senatore Caliendo.

da più parti sono state rappresentate, invece, perplessità sull'inclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 595 del codice penale nel testo dell'articolo 3, sia pure come riformulato con l'emendamento che ho depositato nei giorni scorsi. Credo sia necessario, anzi indispensabile, ribadire che il testo dell'articolo 3, fin dall'originaria formulazione, non lasciava adito ad alcun dubbio interpretativo, per i motivi che ho esposto già ieri. ieri. Lo ribadisco ancora una volta: non era possibile e non era previsto dall'applicazione della nuova normativa alcun aumento di pena nei confronti della diffamazione a mezzo stampa, in quanto, per l'applicabilità del contenuto di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, è necessario quel *quid pluris* che è costituito dall'intento ritorsivo dell'agente.

Nondimeno, come è stato esposto ieri in discussione generale, è anche da considerare che in Commissione giustizia è in corso la discussione

auspico - anzi chiedo - l'approvazione nei tempi più brevi possibili, per mettere fine anche a tutte le discussioni che vi sono state negli ultimi periodi, in quanto esso elimina

D'altro canto, l'espunzione dell'articolo 595 del codice penale dal testo dell'articolo 3 non incide affatto sul contenuto dell'intero disegno di legge, anche in considerazione della marginalità della casistica esaminata, come emerso nel corso delle audizioni: la casistica sulla diffamazione, come atto intimidatorio e di violenza nei confronti degli amministratori locali, è emerso essere un'ipotesi abbastanza marginale e residuale.

con l'emendamento 3.300. Voglio sottolineare che questa decisione è stata assunta anche per fugare qualsiasi perplessità e per evitare che si continuino ad alimentare polemiche, a mio parere - lo ribadisco - totalmente infondate,

Evitando queste polemiche, si cerca anche di favorire una generale condivisione da parte di tutte le forze politiche, così com'è stato fino ad oggi. Si auspica quindi che il provvedimento, anche alla luce degli esiti della discussione, venga approvato, come in precedenza, con una

quegli atti di violenza e di intimidazione non sono diretti soltanto verso la singola persona, ma colpiscono intere comunità, nelle quali, nella maggior parte dei casi, si ha di fronte una buona amministrazione, che evidentemente dà fastidio a qualcuno.

Signora Presidente, per la verità, vedo che continua un dibattito abbastanza surreale. Da un lato il relatore Cucca e coloro che sono intervenuti ieri continuano ad insistere su una cosa assolutamente giusta: la tutela degli amministratori locali, dei sindaci e degli assessori da minacce,

per svolgere la loro funzione. Dopodiché si continua a sottacere che invece questo provvedimento riguarda i parlamentari e i magistrati. Nessuno ancora in quest'Aula mi ha spiegato perché si continua a parlare di amministratori locali, quando invece tutte le norme che introduciamo nel codice, riferite agli amministratori locali, vengono automaticamente estese ai parlamentari e ai magistrati. Ricordo ancora una volta che per i parlamentari

c'è tutta una casistica che sta a testimoniare che, essendo gli stessi magistrati a giudicare, un occhio di riguardo per i loro colleghi, quando si tratta di un conflitto con un giornalista o con un cittadino, ce l'hanno il collega Cucca dice che è emerso dal dibattito di ieri un problema che riguarda

Colleghi senatori, abbiamo portato in Assemblea un provvedimento che aggrava da un terzo alla metà la pena per la diffamazione, quando in Commissione giustizia si sta discutendo, con il consenso generale, di eliminare le pene detentive per il reato di diffamazione. Quindi si proponeva un'aggravante per una fattispecie, estendendola ai parlamentari e ai magistrati, nel caso in cui fossero colpiti da questa campagna ritorsiva e diffamatoria quando, nel contempo, in Commissione si sta andando su posizioni diametralmente opposte.

ai parlamentari e ai magistrati una norma che già nel titolo e in tutti gli interventi dei colleghi è stata motivata dal fatto che una Commissione d'inchiesta ha giustamente rilevato con preoccupazione l'accentuarsi di attentati e intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Non ho sentito nessuno dire

Se lo leggo nei confronti degli amministratori locali, non sono d'accordo con questa affermazione. Se invece leggo quello che sta accadendo, cioè che si vogliono estendere ai parlamentari e ai magistrati un'ulteriore limitazione e un aggravamento di pena per chi si mette nella condizione

alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un provvedimento legislativo. Mi chiedo quindi

o diventa qualcosa che giuridicamente può portare a un processo? Secondo noi, aver esteso ai parlamentari e ai magistrati questa tutela, giusta per un atto amministrativo, per qualcosa di concreto che riguarda gli amministratori locali, è un gravissimo errore.

Signora Presidente, sarò molto sintetico. Noi abbiamo presentato emendamenti che andavano in due direzioni principali: la prima è quella di eliminare il riferimento alla diffamazione, che fosse limitata alla condotta di natura ritorsiva, ma che comunque riteniamo inopportuna per il pericolo di abuso, per le difficoltà interpretative e, sostanzialmente, per un'applicazione che poteva effettivamente prestarsi a una pluralità di interpretazioni non sempre nella direzione che si poteva invece auspicare nell'indicazione di questo reato.

ma una Commissione sulle intimidazioni ai danni dei politici nazionali o locali. Non voglio dire che non si possa discutere dell'argomento, ma mi sembra assolutamente fuori luogo comprendere un'estensione della portata della norma anche al Parlamento nazionale e quindi ai parlamentari.

eccessiva e contraddittoria rispetto al fatto che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse. Quindi aumentiamo la distanza tra parlamentari e cittadini e, soprattutto, apriamo la strada alla possibilità di denunce penali sulla base di questa norma, e non di quelle già esistenti da cinquant'anni che tutelano i parlamentari, rispetto a chi - come vedremo dopo - potrà essere oggetto di atteggiamenti ritorsivi o di chi semplicemente, come abbiamo visto nell'articolo 1, potrà essere colpito se minacciato per ottenere, ostacolare o impedire l'adozione di qualsiasi provvedimento anche legislativo. Io mi domando come si possa inserire nel codice penale un comma che colpisce penalmente un cittadino, un giornalista, un'associazione che minaccia per ottenere, ostacolare o impedire l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, riferito a singoli parlamentari. Mi sembra un altro passo verso la limitazione della libertà. Parlamento ha la mania di dire che vuole depenalizzare, ma poi continua a rendere penalmente colpibili con nuove fattispecie di reato anche condotte che penalmente colpibili non sono mai state o con aggravi di pena o con l'introduzione di nuove figure su cui poi la giurisprudenza dovrà faticare per scoprire quali sono i limiti di applicazione di questa norma. norma. Insisto nel dire che non dobbiamo fare una norma per la casta, una norma di autotutela: noi dobbiamo tutelare gli amministratori locali e non i politici e la politica.

Signora Presidente, condividendo sul punto le osservazioni del senatore Giovanardi, mi corre l'obbligo di fare presente a lui e anche agli altri colleghi dell'Assemblea che se condividiamo l'idea che i parlamentari

che può essere isolata qui ma non lo è nel Paese - per tutelare gli amministratori locali e oppormi a queste norme di autotutela della casta dei parlamentari.

ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

339-*bis*, non si applica in relazione ai componenti delle Assemblee legislative nazionali. Torno sul punto anche in replica al senatore Giovanardi, che evidentemente questa mattina non ha la solita lucidità, nel rappresentare anche a lui che, con questo emendamento, vogliamo esplicitamente escludere i membri delle Assemblee legislative nazionali da questa tutela perché, francamente, misura ultronea, non necessaria, che potrebbe dare adito a polemiche su una tutela della casta parlamentare che vuole difendersi da possibili atteggiamenti di questo tipo.

fare riferimento a delle polemiche, che hanno trovato spazio anche sulla stampa, in cui il senatore Giovanardi addebitava al Movimento 5 Stelle la volontà di mettere un bavaglio alla stampa e di intimidire i giornalisti, sostenendo la necessità di mantenere il reato di diffamazione come aggravante nei casi previsti dall'articolo 339-*bis*. Anche questa è l'unica occasione che abbiamo, come Gruppo politico, per smentire clamorosamente quanto il collega ha sostenuto in maniera un po' proditoria due settimane fa, facendo dei comunicati mirati e infondati. Lo facciamo semplicemente analizzando il testo degli emendamenti emendamenti depositati. Da essi risulta, in maniera paradossale rispetto alle asserzioni del senatore Giovanardi, che lo stesso collega nei suoi emendamenti ha voluto mantenere in diversi casi il reato di diffamazione come aggravante nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti delle categorie protette. Mi riferisco agli emendamenti 3.200 e 3.203, sempre a prima firma Giovanardi, dove addirittura si vogliono escludere le lesioni, le minacce e la violenza privata

Signora Presidente, utilizzo la dichiarazione di voto su questo subemendamento per esprimere il pensiero del mio Gruppo in ordine all'articolo 3 del disegno di legge e al relativo emendamento del relatore. Noi riteniamo che sia l'articolo 3 che l'emendamento del relatore costituiscano un errore tecnico e possano dare luogo ad anomalie interpretative con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 338 del codice penale, così come modificato dall'articolo 1 testé approvato. Perché si dice questo? Nell'articolo 1 che abbiamo approvato puniamo, ai sensi dell'articolo 338, gli atteggiamenti di violenza e di minaccia compiuti anche a causa dell'avvenuto rilascio o adozione di un provvedimento. Siamo in presenza di un reato complesso, cioè sostanzialmente di un reato la cui fattispecie prevede al suo interno un altro reato, sia esso il reato di minaccia, sia esso il reato di violenza.

un reato complesso, che prevede al suo interno altri reati, di violenza e di minaccia, che assumono apprezzabilità penale quando vengano commessi anche a

che, ove fossero commessi all'interno della fattispecie prevista dall'articolo 338, avrebbero una punibilità autonoma e non sarebbe davvero possibile punire due volte lo stesso identico fatto.

posso comprendere che si possa affermare che questi reati possano essere scissi dall'articolo 338 e quindi sostanzialmente, non essendo ad esso collegati, si prevede una possibilità aggravante. Tutto questo sarebbe possibile

Caro senatore Cucca, prendo atto della sua riformulazione che indebolisce, a mio avviso, il testo del suo emendamento quando dice: «a causa del compimento di un atto». un atto». Mi dovete spiegare la ragione per la quale se io compio una minaccia nei confronti di un amministratore locale dopo il rilascio di un provvedimento vengo sanzionato secondo la pena prevista mentre se la compio nei confronti di un amministratore locale a seguito del compimento di un atto che, per ipotesi, è esattamente il rilascio di un provvedimento,

Credo che questi confini non siano chiari e che ciò possa dare corso a notevoli e non indifferenti difficoltà interpretative. E allora, se proprio si vuole immaginare una aggravante diversa per un determinato tipo di reati, dovreste essere molto più chiari nella formulazione, perché quando dite che chiunque commetta reato di minaccia nei confronti di un componente di un consiglio comunale, regionale o quello che è,

Noi riteniamo che questo sia un errore tecnico e che se proprio si voleva inserire un'aggravante, tale aggravante doveva essere scritta

l'articolo 1, cioè la nuova formulazione dell'articolo 338 del codice penale che prevede come reato la violenza o minaccia diretta ad un componente di un corpo politico,

o, se c'è stato un diniego, di ottenere la concessione. Ma l'obiettivo è sempre piegare la volontà dell'amministratore. Quando, invece, si parla di aggravante, si parla di natura ritorsiva perché in tal caso non c'è più questo obiettivo. L'atto si è esaurito. Vi è stata, ad esempio, la demolizione di un immobile abusivo. caso, il titolare o proprietario che si risente di quest'azione, assolutamente legittima dell'amministratore, compie una ritorsione. Egli non ha l'obiettivo di piegare l'amministratore, ma di punirlo a modo suo e reagisce

Presidente, intervengo perché francamente non capisco quale sia lo spirito dell'emendamento Nel nostro sistema il Parlamento e l'esercizio della funzione parlamentare sono particolarmente tutelati, anzi alla libertà di esercizio della funzione parlamentare la Costituzione e i Costituenti dedicarono addirittura la formulazione dell'articolo 68, come peraltro ha ricordato oggi il senatore Giovanardi; quindi, libertà di esercizio della funzione parlamentare come bene e valore dell'ordinamento, tutelato costituzionalmente, che riceve peraltro nel codice penale, come sappiamo di impronta anteriore all'approvazione della Costituzione e alla Repubblica, una tutela specifica che è quella consacrata nell'articolo del quale ci stiamo occupando. Oggi ci troviamo a discutere di un'ipotesi di aggravante per una serie di reati che sono anche particolarmente gravi, perché sono reati di violenza e di danneggiamento. Non c'è più la previsione del reato di diffamazione; è stato un modo con il quale il relatore ha raccolto una serie di obiezioni, a mio avviso, infondate e direi anche piuttosto fragili. Comunque, ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di aggravamento quando questi reati, particolarmente gravi, con contenuto e finalità ritorsiva vengono adottati nei confronti dei rappresentanti di un corpo politico o di un corpo amministrativo. Tutela che l'ordinamento ovviamente prevede in ragione della necessità di assicurare quella libertà di esercizio di funzioni delicatissime del nostro sistema, che sono quelle politiche e giudiziarie,

qualora il fatto sia commesso nei confronti dei rappresentanti delle Assemblee legislative nazionali, a parte il fatto che è palesemente incostituzionale, è del tutto oscura. oscura. Capisco che c'è una delegittimazione della politica, che certamente nel nostro Paese va recuperata, ma pensare che questa delegittimazione investa esclusivamente i rappresentanti delle Assemblee nazionali, al punto che fatti gravi, di natura ritorsiva, commessi nei loro confronti, in loro danno, non debbano vedere la contestazione e l'applicazione dell'aggravante, è un mistero eleusino. Soltanto un modo - lasciatamelo dire - piuttosto pedestre di concepire l'ordinamento e le sue istituzioni, nonché l'equilibrio del sistema e la tutela dei valori costituzionali,

se scorressimo le cronache degli anni, non solo della Repubblica, ma anche del periodo precedente, scopriremmo come invece la tutela rafforzata, penale, un senso l'aveva, l'ha avuto e l'avrebbe avuto qualora fosse stata tenuta nella debita considerazione. Questa esclusione che senso ha, se non quello di una punizione «simbolica»? Probabilmente il reato non verrà contestato, verrà contestato raramente, ma dire che bisogna scrivere che si deve escludere l'applicazione dell'aggravante

del Movimento 5 Stelle, che da una parte inneggia al Parlamento e alla libertà di esercizio della funzione parlamentare e contesta giustamente anche le leggi elettorali, che hanno evitato che si saldasse nel momento dell'elezione il rapporto di rappresentanza tra i cittadini e il Parlamento, e

perché assolutamente in contrasto con il nostro sistema costituzionale, che considera ancora il Parlamento il cuore del sistema e gli appartenenti al Parlamento dotati addirittura mi scuso, ma non accetto lezioni sulla dignità del Parlamento da un componente della maggioranza che sostiene un Governo che non riconosce alcuna dignità a questo Parlamento, con l'abuso della decretazione d'urgenza

proprio per una battuta, essendo il primo firmatario di questo emendamento. Il motivo è sostanziale e l'ha detto la senatrice Finocchiaro: la libertà di esercizio della funzione parlamentare è già tutelata. Non sono parole mie, ma della senatrice. è inoltre un problema di metodo. Come siamo arrivati a definire questo disegno di legge, Presidente? Ci siamo arrivati dopo un anno di lavoro di una Commissione d'inchiesta, costituita dal Senato proprio per indagare sulle intimidazioni ai danni degli amministratori locali; una Commissione d'inchiesta che ha lavorato per un anno e che ha fatto giustamente una serie lunghissima di Senatrice Lo Moro, quanti rappresentanti delle Assemblee legislative nazionali sono stati auditi? Quante giornate, nell'arco di un anno di lavoro della Commissione, sono state dedicate alle intimidazioni ai danni dei politici nazionali? Si è formata la convinzione, all'interno della Commissione, che si stesse andando a operare con un intervento legislativo che avesse una portata di copertura anche dei rappresentanti politici nazionali? Glielo dico io, e mi corregga se sbaglio: zero. È per È per tale ragione che questo emendamento ripristina, credo, anche l'unanimità di convinzione e di determinazione nell'approvare questo provvedimento. All'interno della Commissione c'è stata unanimità e ci può essere unanimità anche in Senato. Sicuramente ci può essere il sostegno anche del Movimento 5 Stelle, espungendo, però, l'applicazione di questo provvedimento anche alla funzione dei parlamentari che, come ha ricordato la senatrice Finocchiaro, è già tutelata.

credo abbia impartito - mi si passi il termine - una lezione di diritto. Piaccia o non piaccia, lo si comprenda o non lo si comprenda, il diritto si ispira a determinate regole, alcune delle quali hanno valenza costituzionale e, come tale, non possono essere bypassate anche per spicciola demagogia. È singolare il ragionamento svolto dal senatore Cappelletti. Poiché la Commissione non si è interessata delle eventuali minacce o violenze nei confronti di parlamentari, ma solo degli amministratori locali, non è necessario inserire nella norma anche i parlamentari. certo dai fenomeni, ma hanno un loro contenuto generale. E pertanto vorrei chiedere al senatore Cappelletti: perché, ad esempio, questa aggravante potrebbe essere rubricata nei confronti del componente di un'assemblea legislativa regionale e non potrebbe, secondo il suo emendamento, essere rubricata nei confronti del componente di un'Assemblea legislativa nazionale?

una tragedia enorme per questo Paese, e se il reato evidentemente non fosse molto diverso dai reati citati nell'emendamento del senatore Cucca

e non leso, che trovò la sua morte dopo giorni e giorni di sequestro, proprio per aver esercitato il suo mandato e le sue funzioni di parlamentare in un determinato modo. E non crede, senatore Cappelletti... che, probabilmente la demagogia che in parte ispira questo suo emendamento non sia una demagogia di poco conto, che evidentemente si scontra con quei principi giuridici che sono stati più volte richiamati? Infine le chiedo, poiché le norme vanno avanti e spesso non muoiono in ragione di modifiche legislative: quando, se mai accadrà, dovesse entrare in vigore la riforma costituzionale e vi dovesse essere il Senato così come lì disegnato, non troverebbe lei strano che il futuro senatore possa godere, in ragione di un'altra qualifica, di questa tutela rafforzata, mentre invece il parlamentare della Camera no? Secondo me - e concludo, signora Presidente - quando si legifera la demagogia va messa da parte bisognerebbe semplicemente fare ragionamenti che abbiano un senso compiuto all'interno di un sistema giuridico, sempre ove il sistema giuridico sia conosciuto. È per questa ragione che, con riferimento solo a questo voto, il Gruppo di Forza Italia voterà contro l'emendamento

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635

nuova finestra") *(M5S)*. L'emendamento 4.0.200 è volto ad istituire l'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

una misura condivisibile, che si può collegare molto bene alla normativa di tutela degli amministratori locali, che stiamo per votare.

lettura: «Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno le modalità» - non di istituzione, perché esiste già - «di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali,

apprezzamento arrivato al punto che il Governo ha deciso di dare attuazione ai lavori di quella Commissione, istituendo prontamente l'Osservatorio. Ci tenevo a dirlo ed è per questo motivo che

locali)* 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: *a)* effettuare il monitoraggio

abbiamo svolto un ottimo lavoro. Ringrazio tutti coloro che insieme a me hanno partecipato a tale lavoro, che ci ha permesso di capire bene le problematiche connesse a questa realtà. Del resto, molti di noi hanno avuto esperienza anche come amministratori locali e chi, come me, è stato direttamente colpito da queste intimidazioni può capire bene il sentimento che prova un amministratore locale

Diventa sempre più difficile per un amministratore locale oggi amministrare sapendo di non essere tutelato. Ormai i sindaci, gli assessori e i consiglieri sono dei veri e propri *front office* e rappresentano lo Stato sul territorio. pongono mano a tutti i problemi più importanti, dalle questioni occupazionali al rilascio delle autorizzazioni: parliamo di autorizzazioni importanti, in molti casi quelle sulle aree demaniali, di fatto sono oggetto di interessi non sempre molto chiari. Quindi, chiunque abbia vissuto questa esperienza sa come questo disegno di legge possa essere un primo importante obiettivo da raggiungere.

riteniamo che ci siano anche tutte le condizioni perché questo provvedimento venga approvato immediatamente. Quindi noi, come Gruppo dei Conservatori e Riformisti, esprimeremo un voto favorevole.

Presidente, colleghi senatori, a una manciata di giorni dallo svolgimento di un rilevante turno di elezioni amministrative oggi siamo chiamati qui in Aula ad approvare un disegno di legge che rappresenta il precipitato di un lavoro importante e necessario compiuto dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Il 5 giugno appena trascorso si è votato non solo in città importanti come Milano, Napoli e Roma ma si è tornato a votare, ad esempio, in Comuni dove i tentacoli della malavita e delle organizzazioni criminali avevano, per così dire, sospeso il tempo e il luogo in cui la democrazia consuma i propri riti delle operazioni elettorali, privando di fatto intere comunità della loro ordinaria rappresentanza elettiva. Il lavoro e lo sforzo compiuto dalla Commissione giunge infatti e fonda le sue stesse ragioni costitutive in un momento nel quale si è andata registrando una vera e propria *escalation* di fenomeni intimidatori nei confronti degli amministratori locali. fenomeni che, come evidenziato nelle audizioni e nelle diverse missioni compiute dalla Commissione stessa, si esplicano in modi eterogenei, si sviluppano con pratiche differenti, vengono attuati e perseguiti tendendo a limitare l'esercizio delle funzioni degli amministratori, a condizionarne le scelte politiche, calpestando e violando quella libertà che è alla base della scelta democratica del nostro Paese. Federazione nazionale della stampa italiana qui a Roma, si è aperta da poco una conferenza stampa di presentazione della Prima marcia nazionale degli amministratori sotto tiro. La marcia è organizzata da Avviso pubblico e si svolgerà in provincia di Reggio Calabria il prossimo 24 giugno. Si tratta di un evento organizzato per la prima volta in Italia ed è la risposta di un sano e vigoroso attivismo che reagisce: si oppone a questo *trend* crescente di minacce, intimidazioni e violenze attuate nei confronti di donne e uomini che, da Nord a Sud, governano le amministrazioni locali, opponendosi agli interessi della criminalità. È questo un fenomeno, infatti, che non segue la classica e atavica dicotomia che vede il nostro Paese spezzato in due, sebbene la maglia nera di questo primato, sia certamente da attribuire, se così possiamo dire, alla Sicilia, alla Puglia e alla Calabria. Il legislatore, occorre darne atto, ha quindi fatto più che bene a fotografare, isolare e bloccare tutte quelle casistiche che rischiavano di non rimanere sanzionabili dal nostro ordinamento. a questo importante sforzo, resta quello ancora fondamentale e non derogabile dell'importante presenza dello Stato nei territori perché gli amministratori locali sono al contempo prima espressione e poi anche terminale diretto della presenza dello Stato nei territori e non possiamo continuare ad assistere a fenomeni, giustificati dal cosiddetto riordino secondo mere logiche di *spending review*, di vera e propria ritirata dello Stato dalle località dai territori che invece necessitano dell'azione preventiva e di deterrenza che appartiene allo Stato. La recrudescenza, infatti, di tali fenomeni intimidatori cova sotto la cenere di una crisi economica e sociale che la criminalità tende a voler cavalcare o volgere ai propri interessi. Occorre, quindi, continuare a combinare politiche diverse che coinvolgano diversi livelli per arrivare finalmente a debellare questa piaga che avvelena un terminale diretto del nostro ordinamento. Tutto il lavoro svolto della Commissione merita dunque un plauso per aver contribuito non solo ad affermare l'autorità dello Stato ma anche a ricercare gli strumenti per attuare la tutela e la difesa di chi è chiamato ad esercitare le funzioni dello Stato, di chi è chiamato a rappresentarlo. Siamo di fronte ad uno sforzo di sintesi e di saggio bilanciamento che fornisce nuovi strumenti di tutela per quanti rappresentano con notevole coraggio la pubblica amministrazione, l'autorità giudiziaria e gli enti locali, al di là dunque dell'ancora perfettibile, a mio avviso, articolo 3, nonostante gli smussamenti cercati con la proposta del relatore. Per tali motivi dichiaro convinto il voto favorevole mio personale e del mio Gruppo.

la vita; ma quante volte la Commissione si è interessata dei parlamentari o dei magistrati? E perché, improvvisamente, le norme a tutela degli amministratori locali esposti vengono estese ai parlamentari e ai magistrati? E come vengono estese? La nostra preoccupazione

chi commette la minaccia. Che cos'è la minaccia? Sono andato a controllare, perché occorre che i colleghi abbiano la consapevolezza di cosa parliamo. Per la Corte di cassazione la minaccia è puntare il dito contro una persona e dirgli: «Te la faccio pagare!» È reato di minaccia

però che anche l'imprenditore a cui bruciano la macchina dovrebbe avere una tutela. Non è chiaro perché il parlamentare debba avere una tutela maggiore

penalmente responsabile. Quello che abbiamo scritto nell'articolo 1 riferito alla legislazione, e cioè colpire chi minaccia persino quando il provvedimento è stato già assunto, vuol dire mettersi su un piano pericoloso che già in passato ha visto norme che sono state poi stravolte nella pratica e hanno causato una restrizione della libertà nel nostro Paese. Queste cose le abbiamo dette e sostenute. Siamo soddisfatti perché almeno sulla diffamazione si è capito che parlare di ritorsione diffamatoria, nel senso che un giornale o un movimento di idee,

il tema principale che stamattina è emerso in quest'Aula ha sostanzialmente una natura tecnica, ovvero il confronto è stato di natura tecnica, sul merito del provvedimento mi pare non vi fossero seri contrasti. Si trattava di stabilire se il disegno di legge fosse stato correttamente immaginato e ideato

Per la verità, il confronto che si è sviluppato, in particolare con le osservazioni proposte dai senatori Palma e Caliendo, a me pare un falso problema, perché

Si è voluta fare un'operazione di chiarificazione per evitare ulteriori differenziazioni o diversi orientamenti sul punto.

che è stato definito l'originalismo, e cioè la rigorosa e limitata possibilità per l'interprete di interpretare la norma. Un'eventuale Un'eventuale cultura di tal genere mi fa venire alla mente addirittura il 533 dopo Cristo, quando Giustiniano promulgò il suo *Digesta*, che, appunto,

Napoleone ebbe a dire, leggendo un commento di un giurista: «Il mio codice è perduto». Per finire, addirittura Hitler immaginava un futuro che emarginasse

La senatrice Lo Moro, con la Commissione d'inchiesta, ha ritenuto di consacrare

venne introdotto nel nostro codice il delitto di atti osceni in luogo pubblico, e quella norma è ancora vigente nel nostro ordinamento. Qualcuno, però, mi deve dire se quello che allora

Palma si lascia andare in argomentazioni squisitamente tecnico-giuridico, che sono apprezzabili, per carità. Chi non riconosce al presidente Palma la capacità di parlare di diritto? però, poi si avvicina alla cultura dell'originalismo, che è stata abbandonata e non ha mai attecchito nel campo del diritto. Ha attecchito di più forse nel campo musicale, dove praticamente l'interpretazione talvolta diventa un qualcosa di filologico.

La nostra volontà di legislatore è stata quella di sanzionare le condotte volte a intimidire e a minacciare e gli atteggiamenti di ritorsione nei confronti di tutti.

nell'illustrare le tesi che contrastavano quanto asserito dal senatore. Io mi limito a fare una considerazione molto più semplice: che differenza esiste tra il legislatore nazionale e il legislatore regionale? cioè, che la norma sia applicabile anche per atti nei confronti del legislatore regionale, non si comprende poi perché si dovrebbe escludere quello nazionale.

squisitamente tecnico, per vederlo applicato al di là dell'orientamento giurisprudenziale già apparso all'orizzonte. È stata fatta pertanto un'operazione di tal genere, apprezzabile.

non può lasciarsi andare e astenersi dal voto, perché si voleva che questa previsione fosse inserita nell'articolo 336 Non mi pare autorevole questa posizione, non l'apprezzo e non ritengo di adeguarmi a un siffatto tipo di orientamento.

ormai, quasi proprio come un virus appestante, si sta sviluppando anche su quei terreni dove non si pensava potesse arrivare. Purtroppo l'intimidazione nei confronti dell'amministratore o dell'organo politico o dell'organo politico è un fenomeno tristemente diffuso, com'è stato rilevato da dati cui ho fatto riferimento nel corso della discussione generale, che riportano numeri effettivamente preoccupanti e inquietanti. Anche se, per certi versi, i dati statistici fanno riferimento ad alcune condotte che possono sembrare tipiche - come il proiettile recapitato in busta, ordigni di tipo esplosivo, lettere minatorie,

la più alta rappresentazione dell'attività politica, se per politica si intende la rappresentanza di un territorio. Il sindaco, oggi, è il vero eroe delle istituzioni,

di minaccia, di diffamazione, di lesioni e di danneggiamento nei confronti di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario in conseguenza del proprio mandato. È ovvio che, nonostante l'esito della

per chi riveste una carica come quella politica, giudiziaria o di un amministratore, quasi che chi va a violare questi corpi politici o amministrativi debba essere punito ancora più severamente. Il Il reato va sempre punito e non deve avere rilievo se viene commesso nei confronti di un politico o meno: siamo tutti uguali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il provvedimento all'esame dell'Assemblea non può che essere valutato con favore da parte di chi si pone al fianco di quegli esponenti politici, di quei pubblici ufficiali e di quei magistrati che ogni giorno, nelle periferie più o meno estreme di questo Paese, danno forza provvidenziale alla nostra democrazia, respingendo le pressioni di nuovi e vecchi potentati criminali. Sempre più spesso, infatti, i singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario sono fatti oggetto di intollerabili atti intimidatori, semplicemente per aver compiuto il proprio dovere al servizio delle istituzioni, per aver preteso il rispetto della legge, per non aver accettato logiche clientelari o scambio di favori. Sono circa 1.265 i sindaci che in Italia subiscono minacce durante lo svolgimento del proprio mandato. Sono presi di mira soprattutto i Comuni con piccola e media densità popolare. Sono dati estrapolati da Avviso pubblico e riportati nella relazione conclusiva approvata nel 2015 dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, della quale ho fatto parte. Le Regioni più colpite sono Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna e Liguria. I numeri potrebbero essere ancora superiori se si considerano gli amministratori che non denunciano per timore di ulteriori ritorsioni. L'Osservatorio nazionale sugli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali, costituito presso il Ministero dell'interno per portare avanti e mettere a frutto il lavoro svolto dalla Commissione di inchiesta, ha completato il monitoraggio delle denunce per tutto il 2014 e ha messo a regime il sistema delle rilevazioni eseguite annualmente ogni 30 giugno e il 31 dicembre tramite le prefetture. L'analisi dei dati sugli atti intimidatori denunciati dal 2013 al 2015 conferma che il fenomeno riguarda tutta l'Italia. Il 2014 segna il 19,4 per cento di denunce in più rispetto al 2013 (da 674 a 805), mentre nel 2015 si registra una flessione del 23,1 per cento rispetto al 2014 (619 denunce). La cronaca quotidiana registra il vasto repertorio delle minacce agli amministratori locali, che vanno dalle aggressioni fisiche o verbali alle lettere minatorie, dagli avvertimenti via telefono o attraverso i *social media* agli incendi di autovetture, dai danneggiamenti di beni personali sino all'uccisione di animali domestici. L'ultimo grave episodio in ordine di tempo è stata l'aggressione armata a Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi, che da anni combatte il malaffare e gli interessi malavitosi relativi all'ottenimento e allo sfruttamento illegale di quei territori e delle risorse pubbliche che a essi sono collegate. L'attacco mafioso a colpi d'arma da fuoco è stato respinto grazie alla professionalità e al coraggio degli uomini della scorta del presidente Antoci, a cui va il nostro sentito ringraziamento. A fronte di questi episodi, le istituzioni non devono far mancare il proprio sostegno concreto e fattivo a chi, per contribuire alla difesa dell'ordine e alla promozione della legalità, subisce minacce o azioni ritorsive. A questo proposito, ancora una volta ricordiamo con soddisfazione la proposta di istituzione di una apposita Commissione d'inchiesta su tale fenomeno, di cui abbiamo apprezzato il lavoro svolto e i risultati prodotti, tra cui il disegno di legge al nostro esame. Un ringraziamento particolare vorrei rivolgere alla senatrice Lo Moro, per il suo impegno e la sua competenza, ma soprattutto per come ha condotto i lavori in Commissione. Allo stesso modo deve essere accolta con grande favore l'iniziativa del Ministero dell'interno che ha portato - come accennato in precedenza - all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sugli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali. Questo organismo, nato nel 2015, si è riunito per la prima volta nello scorso mese di febbraio e ha visto la partecipazione del ministro Alfano, dei vertici del Dicastero e dei rappresentanti degli enti locali, tra cui i presidenti dell'ANCI e dell'Unione delle Province italiane. Oltre al ricordato monitoraggio, le attività dell'Osservatorio, finalizzate a proporre azioni mirate ai territori, riguardano gli approfondimenti sulle cause dei fenomeni intimidatori nelle diverse realtà locali. Tali indagini vengono condotte somministrando un questionario impersonale e indiretto agli amministratori locali per «intercettare» la situazione ambientale e il livello di percezione. La vicinanza dello Stato ai rappresentanti delle istituzioni si concretizza anche con l'attivazione, presso le prefetture, di sezioni provinciali dell'Osservatorio, integrate dai vertici territoriali delle Forze dell'ordine, dagli amministratori locali ed eventualmente, a seconda delle situazioni, da rappresentanti di altre istituzioni e Tali iniziative delle istituzioni sono accompagnate da una decisa azione sul campo da parte delle Forze dell'ordine e dei magistrati, come testimoniato dall'operazione coordinata pochi giorni fa dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, che ha colpito con ventidue ordinanze di misure cautelari proprio una cosca mafiosa operante nella zona dei Nebrodi, dedita alle estorsioni, al traffico e allo spaccio di stupefacenti. A tutto ciò deve corrispondere, tuttavia, un adeguamento della normativa penale, affinché chi combatte ogni giorno la mafia abbia a disposizione strumenti adeguati per reprimere e sanzionare tali condotte. E il disegno di legge in esso è stato disegnato proprio per questo motivo: revisionare il codice penale in modo da innovare le modalità di lotta alla criminalità organizzata e creare nuovi e più efficaci deterrenti contro le violenze ai servitori dello Stato e ai rappresentanti delle istituzioni. Infatti, il disegno di legge fornisce nuovi strumenti di tutela per quanti rappresentano con lodevole coraggio la pubblica amministrazione, l'autorità giudiziaria e gli enti locali, introducendo una opportuna modifica dell'articolo 338 del codice penale, che configura il reato di «violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario», per sanzionare chi si rende autore di tali condotte anche a danno di un singolo rappresentante di queste categorie. Si introduce la possibilità di arresto in flagranza per chi commette tale delitto; si configura quale circostanza aggravante a effetto speciale dei delitti di lesione personale, di violenza privata, di minaccia, di danneggiamento qualora siano commessi come ritorsione contro un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario che adempie al suo mandato, alle sue funzioni o al suo servizio. Infine, si prevede una più efficace salvaguardia dei candidati alle competizioni elettorali locali. Questo provvedimento rappresenta il necessario complemento normativo delle politiche e degli interventi a sostegno delle istituzioni finora descritti. È un disegno di legge ben strutturato, lineare ed efficace, che fornisce agli operatori dello Stato, che si battono sui territori per il contrasto al malaffare di ogni tipo, gli strumenti e le tutele più utili e adeguate. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Area Popolare. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle avrebbe mille motivi per votare favorevolmente a questo disegno di legge. Già nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali i nostri colleghi hanno condiviso, insieme a tutti gli altri membri, la volontà di licenziare un testo che fornisca finalmente delle misure legislative a tutela dei numerosi episodi intimidatori o ritorsivi in danno degli amministratori locali. Infatti, il titolo stesso del disegno di legge pervenuto all'Aula - occorre ricordarlo - parla di disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali. Avremmo motivo di votare favorevolmente anche perché in Commissione giustizia abbiamo

Abbiamo accolto favorevolmente la decisione del relatore e del Governo di espungere il reato di diffamazione tra le ipotesi aggravanti previste dal neo articolo 339-*bis* perché, pur con tutte le considerazioni condivisibili dell'intenzione iniziale, avremmo rischiato comunque di limitare il diritto di critica

soprattutto la modifica dell'articolo 338, cioè la tutela anche dei singoli componenti degli organi collegiali politici e amministrativi in modo che essa sia effettiva per un fenomeno che si va diffondendo sempre più. Peraltro,

argomento che ci mette in difficoltà, che non ha visto la nostra adesione ed è diventato oggetto di attacchi secondo il vecchio mantra della posizione demagogica, riguarda l'estensione dell'aggravante

intimidatorio o ritorsivo nei confronti di parlamentari. Nessun audito ha mai rappresentato questa necessità. E l'esempio fatto dal senatore Palma

di senatori si troverebbero in una posizione differente rispetto ai loro colleghi che rimarrebbero al Consiglio regionale. Insomma, sono tutte osservazioni che ci hanno convinto a ritenere che l'estensione anche ai parlamentari della tutela dell'aggravante per i reati che dovessero subire è priva di necessità concreta. Fossimo davanti a casi simili, non ci asterremmo dal considerare la necessità di questo tipo di tutela. Così non è. Pertanto, pur condividendo l'impianto complessivo, con la modifica dell'articolo 338, e confidando anche che il passaggio parlamentare sia anche più rapido nell'altro ramo del Parlamento, il nostro voto, più per un messaggio politico, sarà di astensione sul provvedimento. proprio per questo aspetto che, pur avendone avuto la possibilità in Aula, con emendamenti che abbiamo proposto, non è stato approvato, ossia quello che estende l'aggravante anche i reati commessi in danno dei parlamentari. Noi dobbiamo concentrare i nostri sforzi su quello che era l'intento iniziale, quello riportato nel titolo stesso del disegno di legge: tutelare i consiglieri comunali, i sindaci, magari anche i consiglieri regionali, i Presidenti delle Regioni che sono oggetto di atti intimidatori o ritorsivi. Occorre fare quello e basterà. Per il resto, per i motivi che spero di aver brevemente illustrato, il voto del Movimento 5 Stelle sarà di astensione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto desidero anche io, come componente della Commissione

che quando c'è una volontà politica, al di là della collocazione di partito, il Parlamento è in grado di legiferare, anche se poi a ciò si è sovrapposto il parere favorevole del Governo. Vorrei anche ricordare che tutto il Gruppo di Forza Italia ha preso parte all'azione della Commissione d'inchiesta e ha dato il proprio sostegno al disegno di legge, tant'è vero che lo stesso è firmato dai componenti della Commissione d'inchiesta del Gruppo di Forza Italia. Quello che si presenta oggi e che si è presentato nella Commissione d'inchiesta è un quadro che era ed è a dir poco allarmante di di questo fenomeno, che mostra una chiara differenziazione sul piano territoriale, sia in relazione al numero degli episodi avvenuti che all'incidenza dei diversi moventi di azioni intimidatorie. È un problema reale e ampiamente sentito dagli amministratori locali, che hanno chiesto, a più riprese e ormai da troppo tempo,

Una delle principali cause del fenomeno delle intimidazioni agli amministratori risiede nel clima di sfiducia, che è sempre più forte, dei cittadini nei confronti delle istituzioni, che è da ricondursi anche ai crescenti problemi economici che il nostro Paese sta ancora, purtroppo, drammaticamente vivendo, così come allo sperpero di denaro pubblico da parte di alcune minoranze di amministratori e di amministrazioni inefficienti, oltre che a fenomeni corruttivi. Allo stesso modo tale fenomeno è dovuto alla paradossale situazione nella quale si trovano a vivere gli amministratori locali, i quali sono investiti di crescenti responsabilità, ma purtroppo sono spesso privati di adeguati poteri e soprattutto di risorse per far fronte ai bisogni dei loro cittadini e dei loro amministrati. I cittadini, infatti, che si trovano di fronte a queste - in alcuni casi - inerzie dello Stato, arrivano a pretendere che siano gli enti locali, che sono le istituzioni più vicine al cittadino, a risolvere tutti i loro problemi. E nei casi in cui nemmeno i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali sono in grado di dare delle risposte concrete, ciò porta inevitabilmente a una crescita della sfiducia da parte dei Negli ultimi quarant'anni sono avvenuti oltre 130 omicidi di amministratori locali. Si ricorda come il periodo peggiore furono gli anni Ottanta, che videro ben 80 morti, in particolare in Sicilia, in Campania e in Calabria. Questo fenomeno purtroppo continua a protrarsi nel tempo. Ancora nel 2013 sono avvenuti gli omicidi di Laura Prati, sindaco di Cardano al Campo (quindi non di un Comune ubicato in Sicilia o in Calabria, ma in alcune delle Regioni

Le Regioni più colpite sono la Sicilia, la Puglia, la Calabria, la Sardegna e la Liguria, mentre in altre Regioni il fenomeno è quasi inesistente, ma incomincia a manifestarsi in alcun Regioni particolarmente avanzate nel tessuto sociale e economico, come la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Vi sono diverse forme di intimidazioni ad amministratori locali che vanno da quelle più gravi come incendi di auto o beni privati, utilizzo di armi da fuoco o ordigni esplosivi, aggressioni fisiche, fino a quelle meno gravi, come le lettere e le telefonate minatorie, che però non vanno in alcun modo sottovalutate perché mettono in luce il clima di paura e di incertezza esistente tra gli amministratori. Vi sono, inoltre, purtroppo, moltissimi casi in cui non vengono denunciati episodi di intimidazione per la paura di possibili ritorsioni e questo incide non soltanto sugli amministratori, ma anche sulle loro famiglie e sui loro cari sulle loro attività di carattere professionale ed aziendale. Questo è il clima in cui vivono le amministrazioni locali. Una quota rilevante delle dimissioni dalla carica è dovuta alle intimidazioni subite. Stiamo parlando di oltre 90 decreti di scioglimento di consigli comunali che hanno come causa intimidazioni o omicidi di amministratori locali. Come detto, il tutto nasce dalla crisi sempre più profonda del rapporto fiduciario tra cittadini ed eletti, e questa crisi si sostanzia

Come Gruppo di Forza Italia avremmo preferito che le modifiche fossero apportate all'articolo 336 e non già all'articolo 338 del codice penale, come avevano sostenuto i colleghi Caliendo e Palma.

Come detto, il fenomeno delle intimidazioni, delle minacce e delle violenze è stato per troppo tempo sottovalutato e trascurato dalla politica. Chi ne ha pagato le conseguenze sono state persone innocenti che hanno visto completamente rovinata la propria vita avendo l'unica colpa di voler svolgere il proprio lavoro, scelti dai propri cittadini, al servizio della comunità. È questo il momento di dire basta: che siano le organizzazioni criminali, la criminalità comune o la semplice prepotenza di chi si ritiene al di sopra della legge e delle istituzioni: tutti devono sapere che lo Stato è oggi più vicino ai propri amministratori, a coloro che hanno scelto di servire i propri cittadini e, in buona sostanza, all'intero Paese. Vorrei fare ora un'ultima considerazione di carattere squisitamente politico:

Per tutte queste motivazioni, il voto di Forza Italia, al di là delle criticità che ho poc'anzi evidenziato, sarà un voto favorevole. Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il mio Capogruppo che mi ha affidato questa dichiarazione di voto e dico subito che non approfitterò di questa occasione per parlare della relazione perché è stata discussa, è stata approvata, ne hanno parlato in tanti e perché oggi siamo davanti ad un disegno di legge da discutere. Rispetto ai risultati della relazione, voglio solo osservare

Generalmente ci si è espressi in termini molto positivi nei confronti degli amministratori locali e ciò, probabilmente, per effetto di posizioni politiche dei vari Gruppi parlamentari, ma anche perché la verifica e i risultati dell'inchiesta hanno prodotto una maggiore sensibilità in tutti noi. Dico questo perché altrimenti non potrei io stessa capire perché, fino a ieri, si ignoravano 132 amministratori uccisi, più 11 parenti, ossia decine e decine di persone che negli ultimi quarant'anni sono morte

vuole. Una prima risposta la devo al collega che mi ha chiesto se durante i lavori della Commissione si è mai parlato in termini generali degli atti intimidatori nei confronti della classe politica.

oppure, molto più opportunamente, intervenire su una norma desueta? Abbiamo verificato sul campo che esistevano norme che astrattamente riecheggiavano e potevano essere applicate, ma ciò non avveniva per un'inappropriatezza Abbiamo sentito parlare sul campo dell'articolo 336 del codice penale e del perché la magistratura che abbiamo interpellato non abbia ritenuto adeguata quella norma. Abbiamo sentito anche fare riferimento a norme diverse da quelle di cui stiamo parlando. Ci sono stati casi in cui sono stati contestati lo *stalking* e le estorsioni perché c'erano i presupposti. estorsioni perché c'erano i presupposti. Parliamo di casi in cui sono stati contestati reati molto gravi. Nella maggior parte dei casi abbiamo però trovato magistratura e Forze dell'ordine

che spesso non hanno collaborato perché la mancanza di strumenti ha creato quella sfiducia anche nella possibilità di intervenire a tutela e con applicazione di una legge vigente che ha prodotto non omertà, ma talvolta silenzio e mancanza di coraggio.

storica, in un'epoca completamente diversa. Noi però non abbiamo riscritto quell'articolo. Probabilmente nell'ambito di una riforma del codice penale andrebbe attualizzato anche il linguaggio. Noi siamo intervenuti per dire che quando c'è un'intimidazione, ad un componente di quel corpo politico, amministrativo e giudiziario, si applicano le stesse pene. Dunque, non siamo intervenuti a creare un nuovo reato, non abbiamo modificato l'entità delle pene, ma abbiamo soltanto reso quella norma direttamente applicabile, a prescindere da qualsiasi tipo di interpretazione. C'è allora allora chi ha sostenuto che c'è una differenza di valutazione tra l'articolo 338, che è modificato in maniera adeguata, e l'aggravante. Credo, come ho cercato di dire prima, che una volta che si fa una scelta di questo genere e che l'amministratore locale viene individuato come componente di un corpo politico (a parte il rilievo immediato che non avrebbe senso distinguere a quale corpo politico, perché i corpi politici sono quelli previsti dalla Costituzione,

e quando non sono applicabili fattispecie di reato più gravi, non avremmo potuto che riferirlo allo stesso concetto di componente di corpo politico.

proprio per la diffamazione diretta ad un corpo politico, amministrativo e giudiziario. Quindi oggi ci stiamo scandalizzando, molto a sproposito, di una cosa che, a prescindere da questa legge, c'è già.

Faccio un riferimento preciso. L'articolo 54 della Costituzione richiede dignità ed onore a chi svolge funzioni pubbliche. Chi svolge funzioni pubbliche è il parlamentare, il sindaco, il consigliere regionale. Non si può distinguere a quale rappresentante

Quando, per esempio, un sindaco viene minacciato per fatti che possono essere ricompresi nell'articolo 338 del codice penale, così come riformulato, saranno possibili le intercettazioni telefoniche e le ordinanze di custodia cautelare.

vogliamo tutelare gli onesti, quelli che fanno correttamente il loro lavoro. Ma ovviamente questi stessi strumenti, utilizzati nei confronti di persone che oneste non sono, finalmente disveleranno le pressioni finalizzate all'intimidazione o alla corruzione, molto prima

apprestata nei confronti di una vittima di un reato e, soprattutto, di una persona che è vittima in quanto rappresenta quel pezzo di Stato che spesso è sul territorio? Perché siamo arrivati a questa incriminazione, se non per la considerazione che queste persone, come tutti noi, quelli che hanno una rappresentanza politica, non rappresentano solo se stessi? La propria macchina è un bene privato e il danneggiamento di una macchina che volete che sia; ma danneggiare e incendiare la macchina a un sindaco sarà pure un'altra cosa, se questo atto

e vorrei condividere con voi la gioia per aver fatto qualcosa di utile, che non risolverà i problemi del territorio, ma che sicuramente potenzierà l'attività di chi deve tutelare la vita democratica dei rappresentanti dei vari territori dei vari territori - e non ho paura di dire - noi compresi. Mi sento, infatti, una persona che, con dignità e onore, svolge un ruolo di rappresentanza politica e se fossi vittima di un reato di questo genere mi sembrerebbe normale essere tutelata. Non è un privilegio essere tutelati, quando si fa il proprio dovere con dignità ed onore, ed è anzi un dovere dello Stato che lo fa,

perché non vi volete prendere la responsabilità di dire che si può fare politica e avere dignità*? (Applausi dai

16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti».

«Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima» (disegno di legge n. 2433). Il disegno di legge n. 2433 presentato e depositato al Senato in data 1º giugno 2016, è accompagnato da 85 plichi, contenenti circa 1.124.960 firme, a sostegno del nostro progetto di legge di iniziativa popolare, stabilendo un *record* per quanto riguarda la quantità di firme e la modalità di raccolta ed evidenziando che i cittadini si attivano su tematiche da loro sentite. avvenuto senza alcun tipo o quasi di pubblicità mediatica convenzionale, ma grazie al passaparola, grazie a migliaia di sindaci, che nei propri Comuni hanno messo a disposizione la modulistica scaricata dal sito dell'Italia dei Valori sulla quale poter apporre la firma, e soprattutto grazie alla volontà dei cittadini di partecipare democraticamente a sottoscrivere una legge che porta in sé una tematica molto sentita e percepita, che tocca la sfera personale di molti. A chiedere un intervento legislativo in materia di legittima difesa sono proprio i cittadini. Non si può passare dalla ragione al torto solo perché ci si difende. Il vero problema non sono le Forze dell'ordine, che si vedono costrette a denunciare, o i giudici che emettono le sentenze; il problema vero è la normativa. Il progetto di legge promosso da Italia dei Valori prevede un inasprimento delle pene da due a sei anni per i ladri e l'introduzione del diritto a difendersi nella propria abitazione, senza quindi rischiare sanzioni, e il divieto di concedere un risarcimento ai malviventi che siano stati danneggiati per legittima difesa. Questa legge non vuole scatenare pistoleri o un *far west* metropolitano; ma sicuramente si rende necessario assicurare più protezione a chi agisce per difendersi. Al momento in Commissione giustizia si sta rivedendo il codice penale e di procedura penale. Parallelamente, alla Camera è tornata in Commissione, per essere nuovamente discussa, un'eventuale revisione dell'articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa, Quindi, auspichiamo che il Ministro competente e i relatori dei provvedimenti in materia penale, sia alla Camera che al Senato, prendano in considerazione quanto scritto nella legge di iniziativa popolare, apportando eventuali correzioni, come richiesto dal disegno

d'Aula sulla delicata questione delle adozioni internazionali, in particolare quelle del Congo. C'è un assunto di partenza ed è il seguente: siamo un Paese che è riuscito a portare via dal Congo numerosi bambini, grazie a un sapiente e sensibile lavoro politico. Proprio questo risultato, però, non può e non deve passare in secondo piano, ma soprattutto rischiare di essere adombrato da non sempre fedeli ricostruzioni di cronaca. Insinuare il dubbio che non ci sia differenza tra gli orfanotrofi di Kinshasa e una scuola di polizia, quale quella di Spinaceto, infatti, è ingiusto e scorretto. A tal proposito riprendo un articolo apparso sul giornale "il Fatto Quotidiano", per circostanziare in maniera più netta quanto ho appena asserito. Il quotidiano in questione, il 2 Giugno 2016 scrive testualmente: «Sono atterrati a Fiumicino alle 5,20 del mattino. Fuori era ancora buio. Salendo sull'aereo pensavano forse di essersi lasciati dietro le spalle la durezza degli orfanotrofi di Kinshasa nei quali hanno vissuto due, tre, cinque anni senza aver mai messo piede fuori. Arriva il giorno della liberazione, ma quello che trovano, come prima accoglienza da cittadini italiani, è un furgone della polizia che li condurrà alla caserma Petri di Spinaceto. In attesa del via libera alla consegna.[...] La cronaca di questo calvario è importante.

fresca di delega, la scorsa settimana ha incontrato una delegazione di genitori in protesta e ha speso parole rassicuranti, ma l'ultimo episodio dimostra che il *lifting* non è bastato: anche stavolta il caos ha regnato sovrano. I bimbi da accogliere con premura sono finiti sui furgoni della polizia, stessa sorte ai genitori. Di criminale, però, c'era solo l'indelicatezza delle autorità». Questo è quanto ha scritto «il Fatto Quotidiano». A questo punto mi chiedo se paragonare le nostre forze di polizia a dei carcerieri che prendono in consegna dei bambini, sottoponendoli a un calvario simile a quello degli orfanotrofi della Repubblica del Congo non sia, *in primis*, ingiusto da parte di chi dovrebbe fare informazione. Permettetemi però di aggiungere che ritengo più scorretto che noi, in quanto eletti come rappresentanti della Nazione, quindi uomini al servizio dello Stato, accettiamo in silenzio che gli uomini di un organo come la Polizia di Stato vengano ingiustamente accusati di mancanza di umanità e di incapacità a gestire una situazione come quella descritta nell'articolo. Inoltre, avevo ricevuto anche una *e-mail* dei genitori adottivi e adottanti in cui era e adottanti mai avremmo potuto pensare che si potesse giungere a tanto nella storia delle adozioni internazionali in Italia. Si è toccato realmente il fondo da parte di pochi genitori, su cui nutriamo molti dubbi, circa anche la loro capacità genitoriale, che hanno ritenuto lecito sbattere i propri figli in un video che alimenta una polemica sterile e inutile contro la gestione degli ingressi dei bambini della Repubblica Democratica del Congo, che più hanno sofferto e stanno soffrendo dall'attesa del ricongiungimento con le proprie famiglie. Così come è avvenuto per tutti i bambini entrati in Italia, fino ad adesso, la scelta è dipesa dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) ed è per questo che restiamo ancora più basiti dalla iniziativa dello *staff* della ministra Boschi di voler accogliere in data 25 maggio i rappresentanti di 4-5 famiglie che si celano dietro il Comitato RDC, rappresentanti» solo «di se stessi». Detto questo, essi concludono dicendo che: «Ci sentiamo offesi da questa notizia come da tante altre notizie cui ci hanno abituato in questi mesi determinati giornali, al soldo di alcuni enti restii alla linea di pulizia avviata dalla vice presidente Silvia Della Monica. Per tutte queste ragioni, in qualità di Coordinamento adozioni pulite, che rappresenta la maggioranza delle famiglie della RDC, riteniamo assurda e riteniamo assurda e offensiva questa iniziativa che di fatto, qualora fosse confermata, rappresenterebbe un voltafaccia clamoroso contro coloro che attendono delle adozioni pulite da questo Governo». Personalmente tifo perché anche gli ultimi 15 bambini che sono in Congo, peraltro in questo momento in condizione di sicurezza a Kinshasa, possano raggiungere i loro genitori adottivi il prima possibile. Credo che a noi non resti altro da fare che cercare la verità, imparare da essa e cercare di difenderla.

in cui versa la città di Terni, in cui anche lei stesso è stato in visita qualche anno fa. La rassegna stampa di questa mattina sulla città di Terni parla di una situazione ambientale

e ancora: «Aria e acqua malate nella conca ternana. L'ARPA conferma: nella Conca ternana aria e acqua malate». Leggo soltanto qualche titolo per farle capire quale sia il livello di allarme presente nella città di Terni.

è quella di diventare città nella quale sperimentare nuove tecniche per il monitoraggio dell'inquinamento, dove studiare gli effetti di anni di distruzione del territorio». Io credo che a queste parole noi dobbiamo rispondere con un grido di riscatto per questa città, anche nel silenzio degli altri parlamentari umbri che invito, se le loro poltrone sono ancora belle calde, a venire qui a prendere la rassegna stampa che passo loro molto volentieri. È notizia di questa mattina un allarme proveniente dalla città di Taranto